Signor Presidente, il Governo attribuisce particolare importanza alla definitiva approvazione in tempi certi di questo provvedimento, che, come noto, prevede interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese, in un momento così delicato per la particolare situazione economica e finanziaria internazionale. Peraltro, tale situazione rende preferibile tenere fermo l'equilibrio raggiunto nel testo approvato dalla Camera e confermato dall'esame in sede referente delle Commissioni finanze e industria del Senato, che voglio qui ringraziare per il lavoro svolto.

nostri lavori. La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione del dibattito sulla questione di fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di incentivi. Per la discussione generale sono stati preannunciati dai Gruppi una decina di interventi, della durata di 10 minuti ciascuno. Pertanto le dichiarazioni di voto finali avranno inizio intorno alle ore 19 e la chiama dei senatori intorno alle ore 20. In relazione ai funerali di Stato dei due soldati italiani morti nell'attentato di due giorni fa in Afghanistan - che avranno luogo domani mattina alle ore 10

stiamo per votare l'ennesima fiducia su un decreto-legge con il quale si è persa ancora una volta l'occasione per dare una risposta alla grave crisi che ha colpito il nostro Paese. Questa fiducia è ancora più pesante delle precedenti perché cade nel momento in cui il Governo annuncia una manovra di oltre 27 miliardi che, a quanto sembra, andrà a colpire, come sempre, i più deboli. Si parla di rinviare i pensionamenti (una piccola iattura, non un sacrificio, secondo il ministro Brunetta), di provvedimenti non meglio precisati sui dipendenti statali, mentre si comincia a parlare di nuovi condoni. La scusa per questa pesante manovra è la Grecia, ma la realtà è che il Governo si nasconde dietro quell'evento drammatico per non ammettere che in questi anni ha taciuto la gravità della situazione dei conti pubblici, negando la crisi. Per agganciare un minimo di ripresa, dovevano essere messi in campo interventi ben più corposi, in materia di ricerca ed innovazione, e più incisivi, per tamponare l'enorme falla che si è aperta dal lato dell'occupazione. Stiamo votando un decreto incentivi che impegna solo 300 milioni di euro su misure minime e che, per arrivare a quella cifra, ha sottratto 50 milioni di euro al credito di imposta sulla ricerca e l'innovazione. Nonostante ciò, è più quello che manca di quello che c'è. Le scarsissime risorse sono state spezzettate in un complesso eterogeneo di misure, anche fantasioso, direi, i cui effetti appaiono minimi, contingenti e sicuramente non strutturali. Si attendevano misure per rilanciare i consumi; siamo invece di fronte ad un decreto *omnibus*, peraltro in formato *mignon*: troppo poche risorse per troppi obiettivi. Sono indicati dieci settori e ben dieci tipologie di beni. Da un lato, si inasprisce la lotta all'evasione fiscale; dall'altro, per fare cassa, si pensa già a provvedimenti di condono. Si spazia dai bottoni alla metro di Parma, dalle gru ai battelli solari sui laghi, dando il senso della casualità, della confusione, delle

diviso al proprio interno anche dopo il dramma della Grecia ed il rischio di *default* di altri Paesi europei. Il Governo è sordo anche sotto un attacco così massiccio da parte della speculazione internazionale, che ha rischiato di mettere in discussione persino il futuro dell'Europa. Ben altro passo deve tenere un Governo per il proprio Paese. Il Partito Democratico ha fatto di tutto, al Senato come già alla Camera, per migliorare questo decreto, assolutamente al di sotto delle necessità del Paese, per incalzare il Governo affinché introducesse norme a favore almeno di alcuni fondamentali settori produttivi, quali - per fare solo un esempio - il turismo, che è del tutto assente, ma anche l'agricoltura, ai cui operatori erano state fatte dal ministro Zaia tante promesse in campagna elettorale (ricordo la questione delle accise sul gasolio). anche all'editoria, alle pubblicazioni dei nostri giornali all'estero. Avevamo limitato gli emendamenti, mantenendo solo quelli più significativi. Ce li siamo visti respingere tutti, senza nemmeno una minima spiegazione da parte del Governo, che ha avallato i pareri negativi delle Commissioni con il solito, laconico, insopportabile aggettivo «conforme», che sembra tanto un buco nero dove sempre più spesso questo Governo si va a nascondere. E quindi ci chiamate all'ennesimo voto di fiducia, che noi non vi accorderemo, perché questo provvedimento è quello che è: uno *spot* elettorale privo di contenuti e di obiettivi, che lascia sulle spalle degli italiani il peso di farcela da soli, siano essi lavoratori o imprenditori, in una bufera i cui esiti sono molto incerti, ma dei quali dovrete inevitabilmente sostenere il peso.

lavorato molto - è ancora il segno di un Governo che ritiene la fiducia come via d'uscita alle sue difficoltà, alla sua naturale e tendenziale sfiducia nel dialogo e nel contributo che il Parlamento può dare. Assistiamo ancora una volta ad un modo frammentario di affrontare la questione economica italiana. Siamo stati fra i più tardivi a riconoscere la crisi la crisi più di un anno fa. Abbiamo attribuito alla crisi economica internazionale scelte di tagli alla scuola e all'università decisi mesi prima, quando ancora non era stata dichiarata la crisi. Oggi la crisi nuovamente rappresentata dalla drammatica situazione della Grecia fa dire al ministro Sacconi: faremo di necessità virtù: come dire che approfitteremo di questa sorta di convincimento, di rassegnazione dei cittadini per poter fare ciò che non abbiamo saputo fare in precedenza. dunque ci troviamo davanti a provvedimenti che di volta in volta vengono estratti fuori dal cappello, dal cilindro senza un disegno organico, una visione complessiva delle emergenze che l'Italia ed il più ampio contesto europeo ed internazionale oggi ci impone. Faccio un esempio: stiamo affrontando nella 7a Commissione il grande tema dell'università. Non la chiamo riforma perché quel disegno di legge non è degno di ricevere questo appellativo. Oggi noi sappiamo, soprattutto dopo Lisbona, che la crescita di un Paese è legata essenzialmente alla sua capacità di investire in ricerca, in formazione, in cultura. Quindi non è soltanto un fatto culturale, ma anche economico. Riconosciamo che la situazione dell'Italia è diversa da quella della Grecia, perché il nostro è un popolo di risparmiatori, e questo sostiene molto anche lo Stato, nel suo debito pubblico; però, ammettiamo tutti quanti che quello che manca all'Italia è una crescita reale, forte, convincente. Ebbene, nonostante questo, si taglia, si taglia soltanto! Come se rincorressimo questo mostro che ci è sempre dinanzi. E non c'è invece un pensiero di lungo periodo sullo sviluppo del Paese. Siamo contro gli sprechi; accettiamo i tagli, quando sono giusti: ma non si può accettare di tagliare sulle aspettative per il futuro di questo Paese, aspettative che ancora costituiscono la nostra speranza. Basti pensare a quello che investono gli altri Paesi in ricerca: i Paesi dell'OCSE sono all'1,3 per cento del prodotto interno lordo mentre noi siamo appena allo 0,8, e si continua a tagliare tranquillamente. In modo particolare voglio affrontare un tema specifico, perché anche questo è un decreto che contiene tutto e il contrario di tutto, per cui non è possibile parlare in modo generale, se non entrando nel merito delle singole disposizioni. Il tema che voglio affrontare è quello contenuto in alcuni emendamenti presentati dai senatori Costa e Vita, ed anche oggetto di un ordine del giorno presentato da illustri colleghi della maggioranza, e riguarda le emittenti locali. Questo è un settore profondamente in crisi,

Il Parlamento, nei confronti di queste realtà importanti per il nostro Paese, ha adottato un atteggiamento a dir poco ambiguo. ambiguo. Sono stati già approvati due ordini del giorno, votati all'unanimità, dalla maggioranza e dall'opposizione, in cui si impegnava il Governo entro il dicembre 2010 dovessero essere ripianati quei fondi che sono stati tagliati.

Inoltre, la finanziaria ha già tagliato quei pochi fondi che erano stati erogati. E allora la volontà è sempre quella di mortificare le realtà locali che spontaneamente producono ed incentivano la democrazia nel nostro Paese. Vorrei intanto ricordare che molte piccole realtà locali di questa nostra Italia, fatta di mille piccole e grandi città, vengono sostenute dalle emittenti locali anche nella pubblicizzazione dei prodotti, nel senso che i piccoli imprenditori o le piccole imprese commerciali, che non hanno la forza e la fortuna di poter entrare nella grande pubblicità, trovano in questi strumenti un importante volano per il proprio sviluppo e la propria sussistenza. Ebbene, si continua penalizzare questo settore; almeno il Governo avesse il coraggio di dire, una volta per sempre, no

Bisogna avere questa onestà. Sono enunciazioni di principio che non vincolano in alcun modo il Governo e dunque sono un momento di produzione nulla del Parlamento. Questa è la verità. Sono settimane che si va avanti con mozioni ed ordini del giorno. Poi non ci si deve lamentare quando il Paese e chi soffia sul Paese per il discredito delle istituzioni presenta il Parlamento come un luogo in cui si lavora poco,

un ordine del giorno appassionato, fatto di argomenti convincenti e persuasivi, ma scritto nella consapevolezza di prendere e di prendersi in giro. giro. Io a questo gioco non posso più far finta di starci e dunque non ci sto più. È necessario svelare le reali volontà. Quindi, chiedo che il Governo assuma una posizione netta,

Non lo dico perché è una battaglia di parte o perché sto facendo anch'io quello che fanno i senatori di maggioranza quando presentano i loro ordini del giorno; dico soltanto che abbiamo la necessità e il dovere di una parola chiara nei confronti di un mondo che non è soltanto quello delle emittenti locali, ma il mondo polverizzato del nostro territorio, che ha diritto a vivere in un tempo in cui la massificazione rischia di distruggere le mille realtà particolari che costituiscono la ricchezza del nostro Paese.

su un provvedimento complesso che avrebbe meritato la discussione di merito siamo alle solite: siamo di fronte ad un Governo che maschera le sue debolezze, le sue contraddizioni, ricorrendo - ormai non si contano più le volte - alla fiducia in modo improprio e con una correzione di fatto della Costituzione materiale del Paese che si vorrebbe peraltro trasferire anche in quella formale. Lo hanno fatto già altri colleghi, ma sembra anche a me doveroso rammentare, Presidente, colleghe e colleghi, che, a causa dell'apposizione della questione di fiducia, e dunque del venir meno degli emendamenti, scompaiono dall'orizzonte temporale - almeno quello a tempi brevi e medi, quelli cioè che attengono alla vita concreta del mondo dell'informazione, che è digitale, veloce e non permette più tempi troppo lunghi - misure che

il tema della diffusione della rete a banda larga. In tutti i Paesi, l'investimento in banda larga è uno degli strumenti anticiclici per così dire essenziali. C'è un piano molto bello del presidente Obama, ma in Paesi anche a noi vicini, dalla Finlandia alla Germania, l'argomento «Internet per tutti», Internet veloce, è quello dentro cui si rimette in movimento anche l'economia materiale. Il paradosso, in fondo, della stagione post-fordista, quella dei beni immateriali, è che anche l'economia immateriale ha bisogno di un volano, attraverso l'incentivo, di fatto, della rete disponibile ai cittadini, giovani meno giovani, ed alle imprese, come grande occasione di evoluzione. La cittadinanza digitale richiede la banda larga in Italia; qualche volta nemmeno c'è quella stretta, di banda, in tante parti del nostro bel Paese.

C'è poi un altro emendamento - ne ha parlato a lungo il collega Procacci, e quindi non mi soffermo sul tema - che riguarda non tanto e non solo l'emittenza radiofonica e televisiva locale, e la radiofonia più in generale, in questo caso, un pezzo dell'economia reale, che ha bisogno soprattutto della varietà locale. D'altro canto, in epoca di federalismo, Presidente, colleghe e colleghi, non possiamo contraddirci ogni volta: una molla per un localismo non banale e non corporativo è dare voce anche alle idee, alla pluralità delle esperienze. Un compito che solo quel tipo di emittenza, oggi, a fronte del «Grande fratello» omologato - che si chiami RAI o Mediaset poco importa - può svolgere. Eppure i tagli più recenti della finanziaria portarono, ancora una volta e più

quel campo ha bisogno, invece, non solo di qualche milione di euro ma, soprattutto, di una convinzione che il nostro mondo politico non ha: questo va detto con assoluta franchezza. franchezza. In questi emendamenti era contenuto anche il ripristino, per l'anno 2010, del Fondo per l'editoria. Non sfuggirà a nessuno di voi che molte testate sono sull'orlo della chiusura. Questo non è più nemmeno un appello, ma una constatazione. ripristinare almeno per un po' questo fondo, quindi, in attesa della tanto conclamata riforma dell'editoria. Noi dell'opposizione da mesi diciamo al sottosegretario Bonaiuti di essere pronti a fare insieme che latita in attesa di Stati generali dell'editoria che, nel frattempo, si sono tenuti in Francia e non ancora in Italia, dove furono annunciati assai prima. Dunque, il Fondo per l'editoria permetterebbe a tante testate *no profit* e non legate al mercato pubblicitario di poter vivere e di continuare a sperare. vi sarebbe stato) un emendamento che eliminava quel bruttissimo decreto interministeriale che ha abolito *tout court* le tariffe postali agevolate. Ottomila fogli oggi sono sul lastrico (dai fogli diocesani a quelli

che rimane davvero, nell'amarezza di non poterlo affrontare insieme, perché so di dire parole condivise da molti colleghi e colleghe della maggioranza. Se ne è parlato

degli editori all'estero, che ha recentemente tenuto un bel convegno qui a Roma, nella sede del CNEL, ci ha spiegato i dati diffusivi e anche il coinvolgimento delle comunità nazionali nei diversi Paesi di tutto il villaggio globale.

così modesta da non farsi comprendere nemmeno in una logica di rigido risparmio, quale quella che il ministro Tremonti evoca sempre.

Sono presenti in tribuna gli studenti della Scuola media statale «Luigi Pirandello» di Bolognetta, in provincia di Palermo, accompagnati dal loro sindaco, dottor Gaspare Greco. A loro rivolgiamo i nostri saluti e il nostro augurio per la loro attività di studio e per la vita del Comune.

La risposta è sempre la stessa: non ci sono i fondi. Forse, se invece di spendere 500 milioni per fare il G8 alla Maddalena avessimo speso i soldi per incentivare il Paese, probabilmente i fondi li avremmo trovati.

ma allora, quale è stato il criterio con cui si è voluto scegliere il settore da incentivare?

Già da due anni sostengo che l'uscita dalla crisi non sarebbe avvenuta prima del 2012, perché i dati relativi alla crescita economica mondiale ci portano a pensare che la

non mi occupo di nautica, visto che in questo Senato troppo spesso credo che ci siano tanti terminali di varie *lobby* del Paese. Forse questo Senato dovrebbe incominciare a pensare di lavorare per il bene del Paese e non per *lobby* del Paese. Nel decreto si prevedono tra l'altro incentivi a sostegno della domanda in particolari settori, tra cui la nautica, dedicato un fondo di 20 milioni, che è suddiviso in due obiettivi: la sostituzione di vecchi motori fuoribordo con quelli di nuova generazione a basso impatto ambientale, per i privati; leggendo questo mi sono molto meravigliato. Cosa è successo? È successo che nel giro di 24 ore i fondi sono terminati. Come si evince dal *Report* sempre del Ministero, 1.023.000 euro sono andati all'incentivo per i fuoribordo e 18.970.000 euro sono andati all'incentivo per gli stampi degli scafi da diporto: 162 interventi. Domando: chi sono questi 162? Per quale motivo si è deciso di dare questo tipo di incentivazione alla nautica da diporto? Di sicuro sarà importante sapere come evolverà l'esame della documentazione fornita dai cantieri per l'acquisto degli stampi. Per ogni domanda non andata a buon fine, si può pensare si può pensare di poter liberare risorse per ritornare a finanziare la parte dei fuoribordo? Queste sono le domande che avremmo posto in una normale discussione, senza la fiducia. Ciò che più stranisce è che in un comparto come quello della cantieristica, che in questo momento nel Paese è fortemente in difficoltà a causa della crisi economica, ci siano abbastanza forze, cioè risorse finanziarie nelle aziende piuttosto che per consolidare il mercato che hanno e i modelli che hanno, e i modelli che hanno, per costruire così tanti stampi in un anno difficile come questo e con prospettive di mercato che sappiamo tutti essere, a breve e medio periodo, molto incerte. Mi lascia molto perplesso anche il fatto che la legge è stata molto precisa e dettagliata con i diportisti e i rivenditori per l'acquisto. Ricordo che avremmo potuto cambiare per ogni stampo almeno 160 motori: quindi, parliamo di almeno 6.000-7.000 motori che avrebbero potuto essere cambiati, con beneficio dei cittadini e con beneficio dell'ambiente. Nel decreto si parla di sconto per l'acquisto di stampi per la laminazione sotto vuoto degli scafi da diporto dotati di flangia perimetrale (tra l'altro, sottolineo che questa è una tecnologia molto complicata che pochi sanno fare), ma non c'è per il cantiere alcun obbligo sui tempi entro i quali deve essere costruito, e neppure una data per l'immissione sul mercato del nuovo modello. Chiedo al Governo, al Sottosegretario qui presente: chi controllerà che tali unità siano davvero prodotte? La mia domanda è volta a sottolineare come ancora una volta si parli di incentivi, si parli di mercato, ma qui non ci sono incentivi per il mercato: ci sono incentivi per pochi fortunati. Ho già presentato un'interrogazione e andremo avanti sulla questione, ma questo è il modo con cui il Governo pensa di poter far crescere il Paese, ancora con delle parti che sono privilegiate e i tanti che vengono sicuramente danneggiati.

dovremmo discutere; sono i temi per il futuro del nostro Paese, per la nostra ripresa. Parliamo di 25-27 miliardi di manovra futura, ma questi 25-27 miliardi nascono anche dalle piccole manovre che si fanno tutti i giorni sui nostri territori, perché se non riusciamo a far partire la nostra economia, il problema sarà - come sappiamo tutti - sulle risorse fiscali. fiscali. Qui non c'è soltanto la necessità di andare a colpire gli evasori, ma c'è anche la necessità di rimettere in moto quel fisco che produce, perché se le aziende non producono, non producono IVA e non producono utili, che sono tutte risorse che vanno al nostro Stato. il ragionamento debba essere molto più ampio. Ancora una volta il confronto ci è stato negato. Ritengo che quest'Assemblea abbia la necessità di parlare di economia. Mi auguro che, quando si parlerà

come un tossicodipendente che non sa rinunciare alla sua droga, il Governo Berlusconi è tornato a porre a questa Camera la

per evitarsi il disturbo della discussione, nonché per lanciare al Paese il sottile messaggio che il Parlamento italiano è un disturbo per il manovratore, un disturbo per un Governo che vuole affermare una idea di sé tutta giocata sull'efficienza, sul tempo rapido, sulla decisione. Noi che stiamo qui tutti giorni sappiamo che non è così, ma il messaggio che si vuole lanciare al Paese è questo. Ci sarebbe da dire che, di fronte ad una dipendenza dalla droga della fiducia, il genitore attento del tossicodipendente Governo dovrebbe essere la maggioranza parlamentare che gli dà o gli nega la fiducia.

il Parlamento stava discutendo con competenza i temi del decreto‑legge sugli incentivi; gli emendamenti erano pochi e selezionati, ed era utile per il Parlamento, ma anche per il Governo, approfondirli, respingere quelli che andavano male, approvare quelli che andavano bene e quelli per i quali magari ci poteva essere una convergenza. il genitore disattento, che siete voi, colleghi della maggioranza - devo dire pochi colleghi della maggioranza che state ascoltando questo dibattito sulla fiducia - ha ancora una volta applaudito applaudito il Governo che viene ad umiliare il Parlamento, perché l'effetto combinato del decreto-legge e del voto di fiducia è l'amputazione della funzione parlamentare.

sul versante delle riforme istituzionali. Il programma elettorale del Partito Democratico, che è quello che verrà riconfermato nell'Assemblea Nazionale di venerdì e sabato, sarà di riformare i nostri regolamenti concedendo al Governo che i suoi disegni di legge vengano approvati entro 60 giorni, che è lo stesso termine

dell'opposizione. Oggi noi siamo costretti a fermare i nostri lavori in quanto la Commissione bilancio è bloccata, perché una maggioranza obbediente ai *diktat* del ministro Tremonti blocca tutto quanto comporta il costo di un euro, senza valutare se quell'euro sia speso bene per il Paese oppure no. C'era tanto da aggiungere, da integrare, da togliere e da introdurre in questo decreto-legge incentivi, che poteva registrare una convergenza tra maggioranza e opposizione. Voglio richiamare una delle pochissime richieste del Partito Democratico.

le famiglie bisognose e per quelle che hanno malati a casa che necessitano di apparati elettromedicali che consumano molta energia elettrica. Nel 2009 abbiamo votato insieme un *bonus* gas sempre per questo tipo di famiglie bisognose. Ci sono però alcune zone dell'Italia dove il gas metano non c'è e questo *bonus* non si applica. Una di queste è la Sardegna che, nella prospettiva di collegarsi ai mercati del gas metano dell'Algeria, avrà probabilmente costruito il suo gasdotto solo dal 2014 in poi. di una proposta semplice, non costava nemmeno molto, sarebbe stata finanziata sulla bolletta elettrica e non se ne sarebbe accorto nessuno: raddoppiare il *bonus* elettricità per le famiglie bisognose della Sardegna (all'incirca 50.000-60.000) che non possono godere del *bonus* metano. Sia ben chiaro, colleghi della maggioranza, senatori del Popolo della Libertà e senatori della Lega che venite in Sardegna a fare la campagna elettorale alle varie fazioni del centrodestra: state votando la fiducia ad un Governo che non accoglie la proposta di equiparare la Sardegna al resto dell'Italia nel trattamento a favore delle famiglie bisognose. Anche questa responsabilità vi state assumendo.

la trentaduesima in 24 mesi, con una media di quasi 1,5 al mese - siano in sintonia con le esigenze del Paese reale,

sistemiche, generate - lo dico ancora una volta - dall'avidità dei banchieri adusi a prosperare sui disastri che hanno in precedenza procurato, avendo anche la pretesa, poi, di proporre ricette per uscire dalla crisi.

va (ricordo anche nella cosiddetta Prima Repubblica quel richiamo «la nave va»;,

il 14 aprile 1912, e la tragedia dell'affondamento di una nave inaffondabile, il Titanic,

sudare per farsi rinnovare il contratto, di quei pensionati che non ce la fanno a vivere; mentre da un'altra parte ci sono i bilanci italiane conseguiti sulla pelle dei consumatori e delle imprese, con la complicità della distratta Banca d'Italia spa (di proprietà delle stesse banche).

questione bancaria, che nessuno vuole affrontare, e che è una questione democratica. Sono dati del Bollettino della Banca d'Italia: - mi riferisco agli ultimi dati - è tornato a crescere il differenziale dei tassi applicati in Italia per prestiti, crediti al consumo e mutui. Per i crediti al consumo vi è un *handicap* di 2,16 punti in più, imposti da questo sistema paramafioso bancario italiano, rispetto alla media europea; per i mutui,

e per un prestito di 30.000 euro rimborsabili in cinque anni (ai quali applichiamo i tassi medi imposti in Italia, pari al 4,74

per il credito al consumo, il differenziale è invece ancora più alto, e per cinque anni devono pagare 368,40 euro l'anno.

nel 2008 sono state assegnate a trattativa privata molte opere per il G8, i cui numeri sono importanti: centinaia e centinaia di milioni di euro. Ci dicevano che queste opere avevano un'importanza e un'urgenza tali da essere sottratte anche al controllo democratico del Parlamento. Parlamento. Leggiamo anche le richieste di rogatorie che sono state presentate dai magistrati di Perugia. Voglio ricordare che se non ci fossero stati Firenze

la *privacy* per i mafiosi, come ha detto l'onorevole Santanché! Quando andiamo a vedere l'ex provveditore ai lavori pubblici che risulta intestatario di un conto presso il Bank Julius Baer di Zurigo grazie al prestanome Roberto Di Mario; quando andiamo a vedere Claudio Rinaldi, e vediamo i nomi, leggiamo gli importi e vediamo questa corruzione, che cosa fate voi, signori del Governo e signori della maggioranza? Piuttosto che dire che il fenomeno della corruzione ha urgenza e che ha la priorità rispetto alle altre cose, se si vuole davvero mettere in collegamento le parole con i fatti, voi assegnate

non avremmo saputo nulla di Fiorani e dei cosiddetti furbetti del quartierino; non avremmo saputo nulla delle inchieste di mafia e degli scandali finanziari che hanno rovinato un milione di risparmiatori per un controvalore di 50 miliardi di euro. bisogna davvero ritornare ad un confronto, se lo si vuole, ma non su queste basi, non mettendo il bavaglio all'informazione.

quei cartelli - con i quali, mi dispiace dirlo, l'attuale Governo va a braccetto - e quei monopoli che non fanno certamente il bene dei consumatori o, ancora, le concessioni,

se farete questo, se si ragiona senza chiedere voti di fiducia, se si ritorna a crescere - perché abbiamo un debito pubblico che grava per 30.000 euro su ognuno dei 60 milioni di abitanti per intervenire, lo possiamo fare insieme. Certamente non condividiamo quelle ricette che voi indicate, non per dare un aiuto alle famiglie, ma per continuare ad aiutare la cricca la cricca degli appalti a farsi i propri affari. Noi non siamo assolutamente favorevoli e difenderemo i diritti e gli interessi della povera gente.

Alle attività edilizie, già attualmente considerate libere ai sensi dell'articolo 6 del codice dell'edilizia del 2001 - vale a dire manutenzione ordinaria, eliminazione di barriere architettoniche e opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo - vengono aggiunte nuove tipologie oggi sottoposte a denuncia d'inizio attività (DIA) che riguardano, in particolare, la movimentazione di terreni in agricoltura e la realizzazione di serre stagionali, nonché, previa comunicazione al Comune via Internet dell'inizio dei lavori, interventi di manutenzione straordinaria, opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, installazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici senza serbatoio di accumulo esterno, interventi in aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. Tutte le citate attività devono comunque osservare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, quelle relative all'efficienza energetica, nonché le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio. Si ritiene che l'osservanza dei regolamenti comunali potrebbe limitare la portata della nuova disposizione e renderla meno efficace, nonostante tale disposizione si inserisca in una normativa - il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 - che si pone al di sopra delle norme e dei regolamenti comunali. Il testo, modificato dalle Commissioni, attribuisce particolare attenzione agli interventi di manutenzione straordinaria, che sarebbero quelli più rilevanti e più diffusi nell'ambito dell'elenco delle attività di cui all'articolo 5. Per tali interventi di manutenzione straordinaria, fermo restando il divieto di intervento sulle parti strutturali dell'edificio, si prevede la comunicazione al Comune dei dati identificativi dell'impresa, di una relazione tecnica e di un progetto a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa e con il committente e asseveri sotto la propria responsabilità che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di titolo abilitativo, tenuto conto che gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano chiaramente interventi all'interno delle singole unità immobiliari che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e che pertanto non potrebbero mai aumentare il numero delle stesse unità immobiliari. Occorrerebbe evitare l'utilizzo di nuove terminologie che potrebbero rivelarsi superflue e pericolose poiché potrebbero generare confusione normativa. Il testo approvato dalla Commissione, inoltre, nel sopprimere la clausola che faceva salve le disposizioni più restrittive della disciplina regionale, prevede che le Regioni a statuto ordinario possano estendere la semplificazione a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti, individuare ulteriori interventi edilizi per i quali è necessario trasmettere al Comune la relazione tecnica ovvero stabilire ulteriori contenuti per la medesima relazione tecnica. Si ritiene una miglioria del testo l'impossibilità per le Regioni di restringere l'applicazione delle norme, anche per assicurare pari opportunità tra i cittadini e tenuto conto che le disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia contenuta nel citato dove si inseriscono le nuove disposizioni, costituiscono principi fondamentali e generali dello Stato cui devono aderire tutte le Regioni. Proprio per lo stesso motivo si nutrono alcune perplessità sulla prevista possibilità per le Regioni di estendere la liberalizzazione edilizia anche su ulteriori interventi, poiché ciò potrà creare una diversa applicazione del codice penale sul territorio nazionale (si ricorda che gli illeciti edilizi sono disciplinati dal codice penale). Si segnala inoltre che alla lettera *c)* del comma 1 occorrerebbe aggiungere l'esclusione dall'attività edilizia libera anche delle attività per la realizzazione dei depositi di stoccaggio di gas e di CO2, accanto alle attività di ricerca di idrocarburi, anche ai fini della chiarezza normativa,

infrastrutture necessarie alla rete di banda larga mobile, con tecnologia UMTS o altre tecnologie, per interventi sugli impianti radioelettrici preesistenti. Si tratta, quindi, delle sole modifiche di impianti preesistenti che, secondo il nuovo testo, possono essere effettuate con la semplice denuncia di inizio attività. Al fine della garanzia di eventuali effetti lesivi sulla salute dei cittadini si prevede che la denuncia resta priva di effetti ove, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, sia intervenuto un provvedimento di diniego da parte dell'ente locale competente ovvero un parere negativo da parte dell'organismo di controllo. Concludo, signor il testo precisa che devono essere comunque rispettate le prescrizioni di cui all'articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche e in particolare del comma 3-*bis* il quale, con riferimento riferimento al completamento della rete di telecomunicazione GSM dedicata alla sicurezza e al controllo del traffico ferroviario, impone il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti unitariamente a livello nazionale dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36. Si ricorda inoltre che attualmente la procedura della denuncia di inizio attività è già prevista per l'installazione di impianti con tecnologia UMTS o altre, con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 watt. Anche la Lega Nord ha presentato un simile emendamento.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, Sottosegretario, il provvedimento in questione, su cui è stata apposta - come veniva ricordato - l'ennesima questione di fiducia, si caratterizza per il contenuto di norme insufficienti nella misura, carenti nella forma, inadeguate nei contenuti, ma anche tardive nei tempi e spesso inopportune nel contesto del provvedimento. Il riferimento principale, se non esclusivo, del mio intervento riguarderà purtroppo soltanto la costituzione del Fondo per le infrastrutture portuali, non avendo sufficiente tempo per parlare, come avrei voluto, delle misure più complessive, da quelle fiscali a quelle inerenti agli incentivi per il sostegno alla domanda di particolari settori economici. Interventi, questi ultimi, davvero inconsistenti, tardivi rispetto all'aggravarsi della crisi e - ciò che più sorprende - senza alcun criterio selettivo rispetto ai soggetti beneficiari, per di più sulla base di insufficienti valutazioni a supporto delle scelte allocative. Chiudo rapidamente su questo aspetto, aggiungendo soltanto che deprecabile è stata anche la confusione generata in queste settimane nei cittadini, prima ancora che nei consumatori, anche soltanto per capire quali fossero le regole del gioco, che hanno destato - come evidenziava in maniera molto precisa e puntuale il senatore Ranucci nel suo intervento - non poche perplessità e sospetti. Aspetto, questo, che dà la cifra dell'improvvisazione con cui è stato confezionato questo decreto, evidentemente motivato da altre finalità (probabilmente non soltanto uno *spot* per le elezioni regionali). Entro subito nel merito delle disposizioni che prevedono l'istituzione del Fondo per le infrastrutture portuali. Voglio subito dire che in sé l'obiettivo avrebbe potuto e dovuto costituire una cosa buona e giusta, perché solo chi se ne occupa da tempo può capire la fame di risorse di questo settore, che da tempo le rivendica, quanto tali fondi siano davvero strategici per lo sviluppo economico del Paese e quanto siano necessari tanto al nostro *export*, quanto all'intercettazione dei traffici, che negli anni a venire probabilmente non saranno così crescenti come fino a qualche anno fa avevamo immaginato. Quindi dispiace ancor di più criticare severamente (avevamo proposto, se fosse stato possibile procedere all'esame, un emendamento soppressivo) un provvedimento verso il quale non solo non ci sarebbe stata ostilità o avversione pregiudiziale, ma che anzi da tempo avevamo invocato, reputandone l'assoluta urgenza. Se ve ne fossero state le condizioni, non avremmo fatto mancare il nostro sostegno, qualora fosse stato necessario o fosse stato richiesto, e comunque il nostro convinto apprezzamento. Il nostro disappunto, quindi, è motivato dal dispiacere per una contrarietà che invece è convinta nel merito e nel metodo. Il provvedimento al nostro esame si caratterizza essenzialmente per l'inconsistenza delle misure rispetto alle necessità riconosciute e note, per la mancanza di organicità e l'aleatorietà del contesto in cui si avanza, assolutamente - mi sia consentito - fuori luogo rispetto al lavoro svolto in questi mesi, con lo stesso Governo, nell'8a Commissione del Senato, estraneo anche alla proposta di legge che - lasciatemelo dire proprio consumata sul tavolo del Consiglio dei ministri (mi riferisco all'autonomia finanziaria dei porti, che è altra cosa rispetto all'istituzione di un Fondo*sui generis,* di un'*una tantum* per le infrastrutture portuali), ma soprattutto per l'ingiustificata e ingiustificabile discrezionalità che ne costituisce la vera cifra. Vede, Vede, Sottosegretario, e vedete, onorevoli colleghi, il principio di discrezionalità, come sappiamo bene, è un aspetto molto delicato, nell'azione di governo, anche quando talvolta si rende necessario per adattare il principio normativo all'interpretazione della realtà; con il rischio, purtroppo assai noto ad ogni latitudine nel nostro Paese, che consente di interpretare la norma per gli amici e di applicarla invece per tutti gli altri. Un rischio che diviene certezza insopportabile quando elementi di intollerabile discrezionalità sono contenuti perfino nella norma stessa, come purtroppo è per il caso di specie. Nella previsione di questo Fondo la discrezionalità sembra costituire il principio unico su cui si informa il provvedimento e la misura in questione. Discrezionalità nelle modalità di revoca di risorse già allocate: non si specifica da cosa deve dipendere la giacenza di fondi non spesi per dar luogo al provvedimento di revoca, sapendo bene che differente è l'inerzia amministrativa dall'impedimento esterno all'ente, come differente è la fattispecie dei vincoli determinati dalle procedure di valutazione dal blocco di spesa, tra l'altro operato precedentemente dallo stesso Governo. Discrezionalità nell'applicabilità perfino della misura, che può consentire al Ministro di attuarla o meno a seconda del proprio umore. Discrezionalità nella riassegnazione dei fondi, legandone la possibilità ad un non meglio specificato parametro di capacità di spesa delle singole autorità portuali, da disciplinare con successivo decreto ministeriale. E soprattutto, la cosa che davvero personalmente trovo più insopportabile e che dà veramente più fastidio è la percezione di una concezione proprietaria delle istituzioni e delle risorse pubbliche, intese come cose di nessuno di cui poter disporre liberamente, perché le circostanze lo consentono. Eloquente in questo senso la revoca del finanziamento alla tramvia di Parma, per 172 milioni (lo ricordava in apertura il nostro relatore), dopo che per almeno un decennio essa è stato il cavallo di battaglia dell'allora assessore alla mobilità, e oggi sindaco di quella città, oggetto contenuto e imposto negli accordi-quadro Stato-Regioni-enti locali, ed oggi oggetto invece di spartizione tra Ministro e sindaco per compensare i reciproci fallimenti. Non è pensabile, e forse non è neppure possibile, che utilizziate una norma di legge per revocare e spartirvi risorse pubbliche vincolate da accordi di programma. Non potete intascarvi risorse che non sono più nella vostra disponibilità. Le risorse di quel territorio devono essere rimodulate con i soggetti artefici di quegli accordi. Politicamente vi state impossessando di una cosa che non è più soltanto vostra. Verrà un giorno che sarete chiamati a renderne conto, politicamente s'intende, come azione scellerata di Governo tanto a livello locale quanto a livello nazionale. L'attuale momento di crisi, peraltro, avrebbe dovuto imporvi a mio avviso, ben altra prudenza e attenzione. Così facendo la vostra condotta non fa altro che avvicinare quel momento di giudizio sulla vostra ormai evidente inconsistente azione di governo.

Sappiamo benissimo che la nostra Costituzione prevede una centralità del ruolo del Parlamento nella scrittura dei testi legislativi: penso, per esempio, all'articolo 72 della Costituzione. Questo Governo, invece, ci sta dimostrando, con un abuso della decretazione d'urgenza, non soltanto per nulla a cuore il ruolo, importantissimo, delle Assemblee legislative, ma soprattutto di avere la necessità di usare lo strumento della decretazione d'urgenza e della fiducia per forzare la programmazione dei lavori e in qualche modo per obbligare la sua maggioranza ad assentire su dei provvedimenti su cui, verosimilmente, se si arrivasse ad un voto ordinario non vi sarebbe Veniamo al merito del provvedimento. Credo che questo decreto sia assolutamente al di sotto delle necessità del Paese e, se mi consente, signor Sottosegretario, certifichi assenza di un'idea di politica economica e di politica industriale, che manca completamente in questi due ultimi anni. Non solo questo provvedimento mette pochissime risorse in campo, ma assegna anche fondi con criteri poco trasparenti e soprattutto realizza una serie di microinterventi, distribuiti in settori che oggettivamente non saranno in grado di rilanciare la nostra economia. Credo che il Governo in questi due anni abbia dimostrato di non avere alcuna idea di che cosa voglia dire una seria politica economica e, all'interno di questa, una seria politica industriale. In Aula e nelle Commissioni non abbiamo mai sentito fare una riflessione approfondita su questi temi, anche perché quando un Governo quando un Governo deve elaborare un disegno di politica economica immagino che debba parlare di piani, risultati, obiettivi e soprattutto di mezzi che mette a disposizione per ottenere tali risultati. Di tutto ciò sinceramente, se non in modo molto frammentario, non abbiamo mai sentito parlare questo Governo. Il ministro Tremonti, peraltro in più occasioni, ha affermato che

di sostegno alla ripresa economica occorra innanzi tutto partire dai consumatori, cioè occorra incentivare la domanda e quindi mettere nelle condizioni i cittadini e le famiglie di incrementare incrementare nuovamente la domanda nel mercato. È quindi evidente che questo obiettivo non si può assolutamente raggiungere con il provvedimento che è all'esame dell'Aula. Le risorse, lo abbiamo già detto e lo hanno detto anche altri colleghi nei loro interventi, sono veramente esigue: 300 milioni di euro di incentivi, oltretutto talmente frammentati lei mi insegna, signor Sottosegretario - da essere una misura assolutamente inadeguata. Soprattutto mi chiedo, e chiedo a lei, signor Sottosegretario, perché nessuno ce lo ha spiegato: con quale criterio si è deciso di sostenere questo o quel settore, senza un disegno complessivo di manovra economica? Credo che sia stata più che altro una scelta lobbistica che il Governo ha ritenuto di fare in favore di questo o quel settore, senza però

molti cittadini italiani che in questo momento, o perché hanno perso il lavoro o perché sono in cassa integrazione, non riescono neanche ad arrivare alla fine del mese per dare sostentamento alle loro famiglie,

270 milioni di euro provengono dalle maggiori entrate che il Governo prevede di incassare attraverso le norme anti evasione. Ora, signor Sottosegretario, il Gruppo dell'Italia dei Valori auspica evidentemente che le norme antievasione

Voglio ancora dire che nell'ambito di questi fondi, complessivamente assolutamente insufficienti, vi è anche una destinazione dei pochi fondi certi del finanziamento dell'industria militare di Fincantieri e di Finmeccanica, mentre tutti i fondi incerti vengono destinati, ad esempio, al fondo per il sostegno alla domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica e di miglioramento della sicurezza sul lavoro. Quindi, i pochi fondi certi contenuti nel provvedimento sono destinati a finanziare, non il miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro, ma l'industria militare. Per concludere, signor Sottosegretario, colleghi della maggioranza, questo provvedimento è inaccettabile in un momento di crisi economica come quello che attraversa il nostro Paese. È una presa in giro per gli italiani ed uno spot elettorale

avrebbe potuto essere migliorato. Invece, ancora una volta si è voluto mortificare il Parlamento ma, soprattutto, mi sia consentito dire che con questo provvedimento si mortificano gli italiani.

e anche oggi in Aula. Questo decreto legge, nel complesso, è un provvedimento poco utile sul piano economico e con costi di attuazione da non sottovalutare. In esso sono contenuti diversi elementi e tanti obiettivi, singolarmente sicuramente condivisibili, per i quali, però, sono state messe a disposizione risorse troppo esigue. Si tratta di un decreto-legge di cui si parlava già nel novembre 2009, approvato dal Consiglio dei ministri poco prima delle elezione regionali, che prevede una durata potenziale fino al 2010. Se il proposito che lo ha ispirato era quello di sostenere il nostro apparato produttivo, sarebbe stato più opportuno intervenire in una fase precedente e meno pesante della congiuntura, nella quale una boccata di ossigeno sarebbe stata

Tra l'altro, già nell'intervento di questa mattina in discussione generale avevo sottolineato quale fosse stata la nostra disponibilità nei confronti del Governo presentando pochissimi emendamenti, proprio per togliere il Governo dall'imbarazzo di di apporre l'ennesima questione di fiducia su un provvedimento che poteva avere sicuramente una diversa portata. Il nostro giudizio negativo di oggi è pertanto aggravato

È difficile sostenere che gli incentivi messi a disposizione con simili misure possano promuovere la crescita del PIL, così come non è facile definire politica economica la somma di microinterventi distribuiti affannosamente nel corso del tempo, che in molti casi non sollecitano nuova domanda, ma consentono solamente di anticipare spese già programmate. Con tali interventi microsettoriali si è persa l'ennesima occasione per inaugurare una politica di ampio respiro. Inoltre - lo ripeto - sono state poche, pochissime le risorse messe a disposizione per perseguire i troppi obiettivi contenuti nel provvedimento

per sostenere una decina di settori dovrebbero risollevare il nostro PIL, che secondo le ultime stime dovrebbe attestarsi allo 0,8

oggi state per approvare in quest'Aula a risollevare le nostre imprese. Purtroppo, o per fortuna, le imprese italiane sono rimaste in piedi perché hanno tirato fuori i loro soldi: dico purtroppo, perché dal Governo avremmo dovuto aspettarci un'azione diversa. A ciò si risponderà, come al solito, che le risorse sono limitate e che bisogna tenere i conti a posto. Anche se corriamo il rischio di essere ripetitivi, quello che noi contestiamo sono i soldi spesi male da questo Governo: sono stati investiti dei soldi per ripianare i bilanci comunali dissestati, mentre ci sono alcuni settori che sono in grado di svolgere una funzione di volano per lo sviluppo e la ripresa che necessitano di nuove risorse. Sul fronte fiscale si reintroducono finalmente strumenti contro l'evasione fiscale; tuttavia, sull'evasione si può e si deve fare di più; questa è sicuramente una prima risposta che il Governo può dare ai problemi di finanza pubblica. Occorre però un intervento più pesante sull'evasione, che,

dell'economia tagli realmente le spese e faccia realmente una lotta all'evasione e ai falsi invalidi e speriamo che queste non rimangano soltanto parole, ma si traducano finalmente in fatti. Abbiamo sperato che alcune proposte emendative di buon senso venissero accolte e che il Governo trovasse, nel corso dell'*iter* parlamentare, risorse adeguate alle condizioni in cui versa attualmente l'economia italiana. Sono condizioni difficili - non confermate da me, bensì dalle principali istituzioni economico-finanziarie - che non consentono certo di fare previsioni rosee sul futuro della nostra economia. Ci saremmo aspettati, quindi, un atteggiamento più disponibile. Alcuni nostri emendamenti riguardavano - per esempio - la rottamazione delle caldaie per riscaldamento e delle macchine agricole,

Anche questa ci sembrava una proposta di buon senso. Abbiamo assistito a sanatorie con rientri importanti di capitali dall'estero ad un tasso ridicolo; prevedere una dilazione per un anno per le imprese in difficoltà nei confronti del fisco con una rateizzazione forse forse sarebbe stato un segnale di vera attenzione nei confronti di quelle aziende che si trovano oggi in difficoltà. Sarebbe più opportuno mostrare attenzione verso quei piccoli e medi imprenditori che hanno investito tutta una vita in risorse per attrezzare una azienda, che stanno vedendo morire ogni giorno e non sanno più dove mettere le mani. Non è stata prestata alcuna attenzione all'imprenditoria femminile, a quelle che sono le piccole imprese familiari

che è stato annunciato alla vigilia delle elezioni regionali in pompa magna, come un decreto‑legge contenente un insieme di incentivi per sostenere la domanda interna. Al contrario, ci siamo poi trovati con risorse scarse e, per di più, sottratte in parte al credito di imposta per l'innovazione, che è proprio quello che chiedono invece le imprese per svilupparsi. Di alcune modifiche introdotte si può sicuramente apprezzare la portata e la *ratio*, ma si tratta di norme che non incidono in modo tangibile e con effetti benefici sulle piccole e medie e medie imprese. Vi è poca, anzi pochissima lungimiranza nel non considerare alcune misure che avrebbero invece prodotto effetti benefici. Il Governo e le istituzioni, purtroppo, non sono stati capaci di trovare soluzioni in grado di sostenere questo momento difficile e di contenere un ulteriore e generale calo dei consumi, con tutto quello che ne deriva. Un'azione di effettiva rivitalizzazione dell'economia italiana avrebbe richiesto una politica incentrata sulla difesa dei diritti e del lavoro, con un più esteso ricorso agli ammortizzatori sociali, necessari per fronteggiare gli effetti delle crisi aziendali. A tal riguardo non possono in questa sede non essere condivise le recenti affermazioni del presidente Napolitano: valorizzare il lavoro, liberarne la potenzialità, riconoscere i diritti. A ciò debbono comunque rivolgersi le politiche economiche e sociali e le tendenze dello sviluppo del nostro Paese. Commissioni del Senato, ma anche in Aula alla Camera, non è passato alcun emendamento, né della maggioranza né dell'opposizione. Molti emendamenti sarebbero stati a costo zero e avrebbero potuto dare un formidabile impulso alle nostre aziende e al sistema Italia. Signor Presidente, concludo affermando che questo provvedimento poteva essere una occasione,

perché appare decisamente insufficiente a risolvere quei problemi della quotidianità che riguardano le famiglie, il lavoro,

a molti invisibili: le piccolissime imprese, le partite IVA, i professionisti, appunto, alla ricerca di una qualche soluzione per la quotidianità.

riguarda anche il metodo; mi sembra si possa definire il metodo della sfiducia reciproca. C'è una maggioranza che non si fida di un dibattito adulto, capace di discernere e di riconoscere proposte costruttive.

«Io mi fido di te, cosa sei disposto a perdere», cantava Jovanotti. E se si fosse disposti a perdere un po' della certezza che si ha ragione soltanto quando si è di più e che quelli che sono di meno hanno sempre torto, potremmo anche aprire su temi di straordinaria importanza, come l'emergenza economica, una fase nuova e un passaggio più interessante e forse più utile. Non so se la fotografia di questa sera e il rito che ci accingiamo a compiere con chiamate, passaggi, no e sì, sia quello che davvero serve al Paese per riconoscersi dentro una presa in carico dei propri governanti. Proprio per questo, quando diremo no, lo diremo anche a questo passaggio, a questo rito, che più che di sfiducia dà l'idea di una rassegnazione, alla quale non vorremmo partecipare. In tal senso il nostro no è un no a cui non ci sentiamo costretti, ma che liberamente scegliamo. *(Applausi

certamente hanno risentito della grave crisi economica internazionale. Tuttavia l'Italia, pur essendo stata colpita dagli effetti della crisi, è riuscita a non farsi travolgere da quest'ultima, grazie anche alla straordinaria capacità di reazione ai cambiamenti del mercato da parte dell'apparato produttivo e alla prudenza dimostrata dalle famiglie, oculate nella gestione dei propri risparmi. Dati economici ci dicono che nel 2010 il tasso di disoccupazione è salito dall'8,6 per cento dello scorso mese all'8,8 per cento, mentre il tasso di inflazione si è attestato intorno all'1,5 Rispetto ad altri Paesi europei potremmo quindi azzardarci a dire che il quadro economico italiano non è tra i peggiori. Il tasso di disoccupazione, infatti, nonostante sia in leggero aumento rispetto agli anni passati rimane tra i più bassi d'Europa. La Francia, ad esempio, è assestata al 10 per cento e la Spagna al 20 per cento. Fin dall'autunno del 2008 il Governo ha adottato diversi decreti per affrontare la crisi economica, dando priorità ad interventi che potessero garantire, da un lato, la tutela dei risparmiatori e delle famiglie e, dall'altro, la tenuta del sistema imprenditoriale del Paese. Alla luce della forte contrazione del reddito e della domanda interna e di fronte alla diminuzione dei livelli occupazionali, sono stati adottati interventi di sostegno alla rete degli ammortizzatori sociali che hanno consentito anche l'attuazione di nuovi programmi di formazione per i per i lavoratori posti in cassa integrazione. Per favorire la nascita di nuove iniziative imprenditoriali è stata anticipata la corresponsione delle indennità di disoccupazione in un'unica soluzione a favore dei lavoratori dipendenti. Parallelamente, per sostenere la crescita e rilanciare la competitività del sistema produttivo, si è proceduto a rifinanziare il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e ad incentivare gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione; misura, quest'ultima, che ha permesso di ridurre il divario accumulato rispetto ad altri Paesi dell'Unione europea. Al riguardo, vorrei fare una breve riflessione sull'opportunità di continuare a garantire, proprio in questa difficile fase di congiuntura economica, le risorse alle imprese, specie quelle più piccole per dimensione, che hanno necessità di dare continuità agli investimenti sulla base di quanto realizzato con l'applicazione della cosiddetta Il rilancio dell'apparato produttivo passa tuttavia attraverso la realizzazione di una semplificazione degli adempimenti burocratici per l'avvio di nuove imprese e al rafforzamento di misure di lotta alla contraffazione e tutela del *made* *in* *Italy*. In quest'ambito è stato introdotto nell'ordinamento un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti, al fine di evidenziare il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e di assicurare la tracciabilità dei prodotti stessi a tutela delle imprese e dei consumatori. Il decreto-legge in esame si inserisce quindi in un quadro più generale di interventi che da tempo sono stati messi in campo dal Governo per uscire dalla crisi e favorire una veloce ripresa. Guardando ai temi di natura industriale, giudichiamo importanti le misure adottate per sostenere alcuni settori strategici per il Paese, primo fra tutti quello Al riguardo, è prevista l'esclusione dell'imposizione del reddito di impresa, nel limite di 70 milioni di euro, del valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, finalizzati alla realizzazione di campionari fatti nell'Unione europea dalle imprese di settore, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 fino al 31 dicembre 2010. Sempre sul tema, durante l'*iter* di esame alla Camera, è stata introdotta una norma, frutto di alcune posizioni espresse fortemente dalla Lega Nord, sulla necessità di tutelare i nostri prodotti dalla sleale concorrenza proveniente dai mercati del Sud-Est asiatico. asiatico. In particolare, è stato istituito un fondo con dotazione di 5 milioni di euro per il 2010 in favore delle imprese che operano nel distretto del tessile, a sostegno del sistema di etichettatura dei prodotti recentemente introdotto con l'approvazione della legge sulla commercializzazione dei prodotti tessili, calzaturieri e della pelletteria. Dico questo solo per rilevare che il Governo si è impegnato ad affrontare e a tentare di risolvere i problemi reali del Paese.

Siamo consapevoli, peraltro, di avere a disposizione risorse ridotte e mirate, ma ci auguriamo che si possa realizzare quanto prima un intervento in questo settore, magari dando la possibilità alle famiglie di poter detrarre dalle tasse i soldi spesi per l'acquisto di mobili per la prima casa.

Le basi esistono e sono concrete. Aspettiamo soltanto di poter cogliere, nel più breve tempo possibile, i frutti delle misure fino ad oggi messe in campo per sostenere la ripresa economica ed avviare il Paese verso una nuova fase di crescita.

non ci convince, perché rappresenta uno spreco di opportunità, perché vengono canalizzate importanti risorse finanziarie su obiettivi inconsistenti e perché, ancora una volta, il Governo e la maggioranza, invocando i tempi di decadenza del decreto stesso, pongono la fiducia, rinunciando a costruire un confronto parlamentare in grado di mettere in evidenza le gravi questioni che abbiamo di fronte. Chi ha seguito il dibattito odierno avrà avuto una sensazione piuttosto strana e surreale: mi perdoneranno i colleghi della maggioranza, i contenuti dei loro interventi sembrano riferiti ad una realtà che non ci appartiene, che non esiste, perché sembrerebbe

Non c'è proporzione, signor Presidente e signor rappresentante del Governo, tra i contenuti di questo decreto e delle posizioni espresse dalla maggioranza e la crisi che il Paese vive; non c'è proporzione, inoltre, tra quanto stiamo qui facendo e quanto fanno altri Parlamenti europei che si cimentano con la drammaticità della crisi. Mentre diciamo questo, prendiamo atto positivamente del fatto che l'attuale maggioranza ha reintrodotto norme cancellate solo due anni fa, quando si è voluto vanificare il lavoro avviato per premiare la fedeltà fiscale, attraverso un meccanismo che avrebbe consentito di abbassare le tasse ai lavoratori e alle imprese che le pagano, mediante la progressiva riduzione dell'evasione fiscale. Prendiamo atto che si reintroducono norme cancellate, sarebbe lungo l'elenco dei provvedimenti approvati in questi venti mesi che sarebbe necessario cancellare e correggere. - mi chiedo - per un Paese, per un Governo e per una maggioranza destrutturare il quadro strategico nazionale per il ciclo di risorse comunitarie 2007-2013, paralizzando l'avvio della spesa delle stesse risorse comunitarie per vari miliardi di euro, rischiando di perdere gran parte di quelle risorse per effetto del meccanismo del disimpegno automatico dettato dalla regola «n+2» o «n+3»? È saggio, in una situazione di grave crisi e di debito pubblico consistente, rinunciare a risorse comunitarie che vanno spese bene per sostenere i processi di crescita e di sviluppo del nostro Paese? Cosa si può dire, poi, degli interventi che hanno frammentato i programmi finanziati con il Fondo aree sottoutilizzate, risorse che erano state programmate per realizzare investimenti al Nord, al Centro e al Sud, esattamente come il quadro strategico nazionale prevedeva e a complemento dei contenuti e delle risorse finanziarie dello stesso? Sono stati distratti miliardi di euro dagli investimenti alla spesa corrente, che continua a crescere, a dispetto di tutti gli annunci e di tutti gli *slogan* di facile consumo. Sono state sottratte risorse alla piccola e media impresa, ai Comuni e alle realtà locali, che avrebbero potuto gestire bene politiche anticiclo. Per questa via sono stati paralizzati gli effetti e gli investimenti sostenibili con il programma interregionale "Energia rinnovabile", che ha una dotazione finanziaria di 2,5 miliardi di euro e il programma per l'attrazione turistica, che ha una dotazione finanziaria di circa 2 miliardi di euro per la stragrande parte del territorio meridionale.

che i 250 milioni di nuove risorse per incentivi a sostegno della domanda per particolari e limitati settori si sarebbero esauriti in poche settimane? Era così complicato capire che quelle misure non avrebbero modificato l'andamento dei consumi e generato una nuova domanda? Era così complicato comprendere che quelle risorse non avrebbero determinato un fecondo rendimento di politiche pubbliche necessarie in questo momento? Il rendimento di quelle misure è pari allo zero.

per sostenere ricerca ed investimenti nei settori dell'energia rinnovabile e del ciclo della combustione, delle scienze della vita, del *made in Italy* o della mobilità sostenibile, non avremmo forse potenziato lo sforzo che interi territori stanno sostenendo per non arrendersi alla crisi? Era così complicato ragionare in questi termini ed è così difficile aprirsi ad un dibattito, ad un confronto parlamentare, in grado di discriminare

che il Governo e la maggioranza abbiano una ricetta standard per affrontare le situazioni di difficoltà e per annunciare una volontà di contenimento del debito pubblico: agire sui pensionati, sui dipendenti pubblici e sulle piccole imprese, alle quali imporre nuovi e pesanti sacrifici. Quella ricetta non ci porta lontano e determina un processo di attenuazione degli sforzi,

comprendere che, ad esempio, attraverso misure messe in campo pochi anni fa, attraverso il credito d'imposta per l'efficienza ed il risparmio energetico,

determinando una crescita di fatturato e di gettito fiscale, creando migliaia di posti di lavoro, o salvando gran parte di quelli che purtroppo stiamo perdendo? La situazione è complicata, non si può rinviare oltre un dibattito serio, approfondito. Si rende a nostro parere urgente affrontare la crisi; è necessario guardare in faccia la realtà, anche per giocare da protagonisti in Europa, ove si assumono decisioni importanti. È necessario giocare un ruolo in Europa per non subire le misure che altri Paesi decideranno per salvare l'euro e per contenere questa situazione di grave drammaticità che stiamo vivendo. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, vogliamo chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di recarsi in Parlamento e di raccontare al Paese la verità sui conti pubblici, di spiegare al Paese qual è la strategia che si intende mettere in campo per uscire dalla crisi. Non serve mettere la testa sotto la sabbia: i nodi, prima o poi, vengono al pettine. Non c'è più tempo da perdere, non c'è la possibilità di aspettare che la tempesta passi. Ci vorranno quindici anni per recuperare le perdite subite, se si tornasse a crescere come prima della recessione. Servono scelte strategiche per far ripartire il Paese a tassi più sostenuti. Il nostro Paese ha già dato prova in altre circostanze di grande forza, di grande slancio e generosità ed ha saputo raggiungere grandi risultati, quando gli obiettivi erano chiari e condivisi, quando - in una parola - era chiaro quale fosse l'interesse nazionale. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, il Governo e la maggioranza decidano finalmente di fare la propria.

il provvedimento d'urgenza all'esame del Senato rappresenta un ulteriore tassello dell'insieme degli interventi che il Governo Berlusconi ha adottato negli ultimi mesi per affrontare con forza l'attuale crisi economica. Il decreto-legge costituisce infatti l'ultima delle misure varate dall'Esecutivo, che fin dall'inizio della crisi - è opportuno ricordarlo - è intervenuto con forza per tutelare prima di tutto i risparmiatori, per cercare di evitare strette creditizie alle imprese e alle famiglie, per rilanciare i consumi attraverso incentivi di sostegno alla domanda. La crisi finanziaria, scoppiata negli Stati Uniti e aggravata dalla situazione economica di alcuni Paesi europei, come la Grecia, è intervenuta in un momento in cui gli indicatori macroeconomici e congiunturali testimoniavano una crescita in forte rallentamento. I mutamenti socioeconomici degli ultimi anni hanno infine amplificato gli effetti della crisi. Tuttavia, l'Italia, pur essendo stata colpita duramente, non è stata travolta. Le principali istituzioni economiche internazionali, dal Fondo monetario all'OCSE, hanno assicurato proprio in questi giorni che l'economia italiana è solida e anzi hanno messo in luce come la crescita che si sta registrando risulta superiore alle principali economie occidentali, che - a parte la Germania - stanno risentendo in misura maggiore della crisi rispetto al nostro Paese. La struttura del sistema industriale, basato su una rete di piccole e medie imprese, la capitalizzazione del sistema creditizio, la forte indole al risparmio privato da parte degli italiani hanno consentito e stanno consentendo al sistema Paese di reggere. Il tasso di disoccupazione, nonostante sia risultato in aumento rispetto agli anni scorsi, si attesta comunque tra i più bassi in Europa e nell'intero Occidente. I colleghi di quest'Aula ricorderanno che il Governo è intervenuto più volte con una serie di decreti, mandando dei precisi segnali ai mercati sulla volontà di tutelare i risparmiatori, di salvaguardare la stabilità del sistema bancario e finanziario, di ampliare gli strumenti a disposizione dello Stato per entrare nel capitale delle banche e di far ripartire i consumi, affrontando di petto la forte contrazione della domanda a livello interno e internazionale. Il Governo inoltre - è importante ricordarlo - è intervenuto fornendo i dovuti mezzi finanziari per assicurare un robusto sistema di ammortizzatori sociali con l'estensione della cassa integrazione anche a settori come quello dell'artigianato che in passato non ne avevano mai potuto godere. Il decreto sul quale il Senato è chiamato ad esprimersi si inserisce quindi in questo contesto di difficoltà oggettive, legate agli scenari internazionali, e proprio per questo, lo stanziamento delle risorse che alcuni hanno considerato troppo esigue costituirà un contributo comunque rilevante per i consumatori e per le imprese. Il decreto contiene una parte di normativa fiscale non trascurabile, in linea con le scelte già adottate dal Governo: detassazione del lavoro straordinario, misure per favorire le piccole e medie imprese, semplificazione delle procedure per il pagamento dell'IVA, rivalutazione degli immobili iscritti a bilancio a fronte del pagamento di un'imposta sostitutiva. Tutto questo nell'ottica di un'azione complessiva di contrasto all'evasione fiscale, anche attraverso la repressione dei fenomeni delle frodi carosello consumate in Paesi esteri. È tuttavia sulle parti relative ai settori industriali che voglio concentrare l'attenzione di quest'Aula a partire proprio dalle norme a favore del comparto tessile. Il decreto prevede ad esempio l'esclusione dall'imposizione del reddito d'impresa del valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e sviluppo, precompetitivo, finalizzati alla realizzazione di campionari prodotti nell'ambito dell'Unione europea. Questa misura è chiaramente volta a premiare tutte quelle imprese che decideranno di continuare ad investire in Italia e in Europa. Si tratta di un ulteriore incentivo per le piccole e medie imprese, legate al territorio che decidono di puntare sulla qualità dei prodotti *made in Italy* che sono il fiore all'occhiello del nostro Paese. Gli scenari della globalizzazione che ormai noto consentono oggi di ricorrere alla manodopera a basso costo nei nuovi Paesi emergenti come la Cina, dove tuttavia non vengono quasi mai garantiti e tutelati i diritti dei lavoratori. Per questo, il Governo ha deciso con forza di appoggiare tutte le realtà imprenditoriali che decidano di mantenere i propri investimenti in Italia, garantendo i livelli occupazionali negli stabilimenti italiani. Così è stato con il disegno di legge sulla tutela del *made in Italy*, fortemente richiesto dal mondo delle piccole e medie imprese, e che permette di premiare chi con sacrificio ha deciso di produrre in Italia, valorizzando quelle professionalità e quelle competenze che il resto dell'Europa e del mondo ci invidia. Bisogna sottolineare inoltre che il provvedimento contiene una serie di incentivi per l'acquisto di prodotti che consentono un risparmio energetico che si rivolge a tutte quelle imprese che decideranno di puntare maggiormente sull'efficienza energetica. Anche questi interventi si collocano nel solco dell'azione intrapresa dal Governo in campo energetico, attraverso l'approvazione delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e l'avvio di un percorso che riporterà l'Italia alla produzione di energia elettrica di fonte nucleare. Tutto questo permetterà al Paese nel corso dei prossimi anni di vedere sensibilmente ridotti i costi dell'energia elettrica che le famiglie e le imprese devono sopportare in misura maggiore rispetto agli altri Paesi europei. Il provvedimento quindi, onorevoli colleghi, continua sulla scia del percorso avviato dal Governo Berlusconi, il Governo del fare, attraverso una seria lotta all'evasione fiscale, con un pacchetto di misure di aiuto alle famiglie ed alle imprese, mediante il sostegno alla domanda, di attenzione nei confronti del mondo del lavoro, con particolare riguardo a coloro che si trovano in situazioni di difficoltà. il Gruppo del PdL darà convintamente il proprio voto di fiducia al Governo su un provvedimento che - ricordo - è stato trasmesso al Senato dalla Camera solamente pochi giorni fa e sul quale era inevitabile il ricorso alla fiducia per garantirne la pronta conversione in legge. È un provvedimento strategico per l'azione del Governo che, insieme agli altri già varati dall'Esecutivo Berlusconi, consentirà un rilancio del Paese a livello interno ed internazionale ed una rinnovata fiducia di tutti gli italiani, dando quello slancio necessario per lasciarsi finalmente alle spalle la crisi economica.

di conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.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 Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza. I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza. Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

Giordano, Giovanardi, Giuliano, Gramazio,

Marini, Marino Ignazio,